apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Ministro, l'amministrazione della giustizia è stata penalizzata per oltre due decenni dal mancato *turnover* del personale e dall'accrescersi delle scoperture che hanno raggiunto la cifra di circa 9.000 unità. Considerato che questo disinvestimento nell'amministrazione giudiziaria influisce in maniera determinate sul servizio giustizia e sui tempi di risposta alle domande di cittadini ed istituzioni, dando atto a questo Governo che, sin dal suo insediamento, ha per la prima volta invertito questa tendenza attraverso l'immissione di nuovo personale in mobilità, proveniente dalle Provincie e dagli enti in esubero, grazie allo stanziamento di nuove risorse per l'efficienza del sistema giudiziario; considerato che questo sforzo ha consentito di rispondere sia ad un problema dell'amministrazione giudiziaria sia a quello di tanti lavoratori in esubero nelle loro amministrazioni, si chiede quali ulteriori misure si intenda adottare per potenziare gli organici del personale amministrativo, in modo particolare in quelle aree del Paese che soffrono le scoperture maggiori, come il Veneto (cito ad esempio le assenze del personale amministrativo del tribunale di Vicenza e della procura competente su processi ed azioni conseguenti alla crisi della Banca popolare di Vicenza, che ammontano a circa il 25 per cento dell'organico). Si chiede inoltre come si intenda affrontare il tema della riqualificazione del personale amministrativo della giustizia, altra questione vivamente sentita dall'intero mondo della giustizia.

Le chiedo quali provvedimenti intenda adottare perché, dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si è verificato un ritardo nella celebrazione dei processi in alcuni uffici. quindi ricalibrata la situazione, tenuto conto anche del blocco del *turnover* tra uffici e uffici. Probabilmente questo porterebbe anche a risolvere la situazione della corte di appello di Napoli, cui lei ha fatto riferimento negli ultimi giorni. Le chiedo inoltre se non abbia intenzione di introdurre per legge la sezione tributaria della Corte di cassazione, perché significherebbe incidere fortemente sulla funzionalità della Corte, tenuto conto che un terzo dell'intero contenzioso civile riguarda proprio la sezione tributaria, mentre gli altri due terzi sono ripartiti tra le altre cinque sezioni. Introdurla per legge significherebbe dotare la sezione di un numero sufficiente di magistrati, così come avvenne per la sezione lavoro. GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Ministro della giustizia, a nome del Movimento 5 Stelle chiediamo di conoscere quali siano le linee guida del Governo, in particolare del suo Ministero, per il contrasto alla criminalità organizzata, in particolare sotto il profilo del numero degli organici dei magistrati dei tribunali di prima linea. In particolare, con la Commissione antimafia, abbiamo rilevato una situazione gravissima a Reggio Calabria, dove sono pendenti quasi un migliaio di richieste cautelari, che non vengono esaminate per carenza di gip. Ma questa situazione è presente in parecchi tribunali che sono esposti in prima linea nella lotta alla mafia. Chiediamo - come ha fatto anche il presidente della sezione gip di Reggio Calabria - se non sia necessario addirittura un intervento, com'è stato fatto per esempio per Expo, per smaltire la gran mole di lavoro e soprattutto per non vanificarla. La seconda questione riguarda proprio la soppressione della corte d'appello di Reggio Calabria, che riteniamo essere un danno nel contrasto alla criminalità organizzata. Vorremmo conoscere la posizione del Governo sotto questo profilo. Da ultimo, per quanto riguarda Napoli, non ci sono soltanto i provvedimenti richiesti dalla procura che pendono nei vari tribunali, ma

è evidente che il sistema giudiziario italiano è caratterizzato dalla lunghezza dei tempi dei processi e da un eccessivo carico di lavoro delle corti giudiziarie e, in modo più specifico, da difficoltà legate alla materia dei minori e della famiglia, e della famiglia, cui da più parti, ormai, si avverte la necessità di assicurare concentrazione e effettività di tutela dei minori, con un modello processuale unico e un giudice specializzato. Un tribunale, un ufficio autonomo di procura che accorpino in sé le competenze in materia di persone e famiglie minorenni.

La considerazione comune è che la giustizia minorile italiana sia un patrimonio inestimabile, in quanto mira a produrre risposte adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minore, la cui tutela e riabilitazione ne sono il presupposto e la finalità principale. A tali principi si ispira anche l'Europa, che recentemente ha approvato una direttiva sulle garanzie procedurali per i minori penalmente indagati, che assume esattamente i valori ai quali si ispira il nostro ordinamento. In data 10 marzo la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge che prevede la soppressione dei tribunali per i minorenni e gli uffici del pubblico ministero presso i suddetti tribunali,

dalle Camere, dall'altro ci preoccupa l'autonomia dell'organo giudiziario e la specializzazione, in particolare per le procure e per la loro funzione di prevenzione. Si chiede se il Governo intenda favorire la creazione di un tribunale e un ufficio autonomo di procura che le competenze in materia di persone, famiglia e minorenni, mantenendo e valorizzando, anche attraverso la riserva di esclusività delle funzioni, le competenze e la specializzazione del settore nell'esclusivo interesse del minore. BARANI *(AL-A)*. Signor Ministro, alla luce delle indubbie lungaggini giudiziarie di cui il Paese sembra soffrire in maniera ormai atavica e che tanti danni causano in termini finanche economici, oltre che in materia squisitamente di giustizia, considerata la mancanza di personale - come molti miei colleghi hanno testé detto - presso gli uffici giudiziari, da più parti oggetto di denuncia in riferimento alla lunga durata dei processi (finanche la Corte di giustizia europea ce lo ripete continuamente), ritenuto che tale esponenziale dilatazione dei tempi relativi alla durata dei procedimenti giudiziari, da un lato, è causa di ulteriore calvario per quanti verranno poi giudicati innocenti e, dall'altro, rischia di non garantire la certezza della pena per chi effettivamente è reo, le chiediamo come Gruppo come si intenda procedere al fine di ottimizzare un settore cardine del Paese e se il recente previsto accorpamento degli uffici giudiziari non rischi di rallentare ulteriormente la macchina della giustizia. Signor Ministro, non vorrà mica accorpare il tribunale di Massa Carrara con quello di Lucca, e così tanti altri tribunali in Italia? Sarebbe uno scempio. Noi non glielo permetteremo.

del tribunale di Vicenza, dove c'è una scopertura di organico del personale di cancelleria che ha raggiunto livelli al limite del collasso, una scopertura recentemente arrivata al 25 per cento. Si tenga presente che, nonostante sia stato previsto l'arrivo di nuovi magistrati,

in corso sulla Banca popolare di Vicenza: un grosso filone investigativo che richiede non solo pubblici ministeri, ma anche e soprattutto personale di cancelleria, in modo da poter svolgere questi processi. Per questa ragione le chiediamo quali possano essere i provvedimenti per la ricostituzione dell'organico di tutti gli operatori giudiziari al fine di consentire alle cancellerie del tribunale di Vicenza di funzionare in modo efficiente. DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Ministro, il suo Governo è intervenuto a riorganizzare gli uffici giudiziari di primo grado tramite la soppressione di 220 sezioni distaccate di tribunale, con relative procure, e ben 667 uffici del giudice di pace. Questo intervento di razionalizzazione ha determinato ulteriori gravi aspetti di criticità rispetto alle carenze di organico del personale amministrativo. Non solo: è emerso un ulteriore aspetto problematico connesso allo stato dell'edilizia giudiziaria spesso, già prima della riforma, insufficiente a gestire affari e personale e dunque ancor più in sofferenza per l'ulteriore carico rappresentato dai relativi accorpamenti, determinando un aumento delle udienze e il necessario spostamento di molte di esse a orari pomeridiani. Altro elemento conseguito alla citata riorganizzazione concerne la nota carenza di organico dei magistrati, che ha determinato problemi relativi alle incompatibilità nella trattazione dei processi, la necessità di rinnovazione di atti nel dibattimento con riguardo a giudici trasferiti e il conseguente sovraccarico dei ruoli e il rallentamento della macchina giudiziaria. Tutto ciò ha determinato un notevole allentamento del fondamentale criterio di prossimità, allontanando il cittadino utente dal servizio giustizia, con le inevitabili e nette prese di posizione dell'avvocatura, concretizzatesi in scioperi Dal momento che il Ministero della giustizia ha istituito una commissione di studio, la commissione Vietti, volta a elaborare un disegno di legge delega, il mio Gruppo chiede di sapere quali criteri oggettivi verranno utilizzati per il riordino delle sedi di corte d'appello, tenuto conto degli elementi di criticità già evidenziati nella precedente riorganizzazione Grazie

Signor Presidente, il recupero dell'efficienza degli uffici giudiziari è stato al centro della nostra azione sin dal momento dell'insediamento del Governo. Devo dire che mi viene bene percorrere il filo logico delle vostre domande partendo da quella che è stata posta da ultimo, cioè cosa succede in ordine all'edilizia giudiziaria all'indomani degli accorpamenti. degli accorpamenti. Con la ristrutturazione, che in verità rappresenta l'esercizio di una delega di una legge di stabilità di qualche anno fa, abbiamo prodotto l'accorpamento di una serie di uffici giudiziari, riducendo di circa il 50 per cento l'edilizia utilizzata dal Ministero del giustizia sul territorio. A fronte di questa riduzione consistente abbiamo

complessivamente ha risanato un quadro in cui molti sprechi si erano determinati a causa di un meccanismo che faceva sì che l'ente che spendeva non era lo stesso

in seguito alla soppressione delle Province, o meglio alla riforma delle Province, ci è stato chiesto - credo giustamente - di utilizzare prima i dipendenti delle Province che si trovavano in esubero. così registrato un passaggio di alcune centinaia di unità, meno però di quelle che si aspettavano, tanto che ieri

per dipendenti di cancelleria, dando così una risposta che considero significativa, anche se non ancora sufficiente rispetto all'insieme delle scoperture che si sono venute a determinare. Nel corso di questo stesso periodo abbiamo avviato un percorso di riqualificazione del personale che non vedeva analoghi processi dalla fine degli anni

mobilità e nuove assunzioni a riqualificazioni, perché questo prescrive la legge. Quindi, una volta conclusa la mobilità e avviato il concorso, potremo procedere alla riqualificazione di altri dipendenti. Per quanto riguarda le singole domande che sono state poste e che mi sembrava giusto inserire in un quadro di carattere generale, rispondo che gli uffici generali di Vicenza hanno urgenza di recuperare le risorse umane da destinare all'efficace funzionamento della macchina giudiziaria, posto che l'ufficio presenta una percentuale di scopertura del 22,48 per cento rispetto alla media nazionale del 21,72 per cento (quindi si discosta relativamente poco) e a quella distrettuale del 19,36 Grazie agli interventi già avviati di mobilità sono state immesse in servizio sei unità ed è ancora possibile ricorrere allo scorrimento della graduatoria esistente per la copertura di un ulteriore posto. Inoltre, a seguito della condivisione della graduatoria di un concorso bandito dall'Istituto per il commercio estero, è stato possibile coprire due posti di funzionario ed è ancora in corso la procedura di scorrimento per la copertura di un'ulteriore posizione. Nel 2015 è stata altresì assunta un'unità appartenente a categorie protette. Con riguardo all'ulteriore procedura in corso, secondo le previsioni della legge di stabilità, altre unità potranno essere assegnate all'ufficio attraverso il portale gestito dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la Provincia di Vicenza sono state inoltre individuate tredici unità. Infine, sono stati assegnati otto tirocinanti all'ufficio per il processo di Vicenza, sei dei quali sono già operativi. Con riferimento, invece, alle questioni poste dal dal senatore Giarrusso, riferisco che la percentuale di scopertura del personale amministrativo del tribunale di Napoli è pari al 28,14, destinata a diminuire all'esito della definizione del bando di mobilità. Con riferimento alle dotazioni degli uffici, comunico che il Ministero ha svolto una complessiva ricognizione delle esigenze degli uffici su tutto il territorio e sta ridefinendo le piante organiche della magistratura, con conseguenze naturalmente anche sul personale amministrativo. Per quanto riguarda i cosiddetti tribunali di prima linea, il tribunale di Reggio Calabria, secondo la proposta che stiamo per avanzare al Consiglio superiore della magistratura, prevedrebbe un incremento nella pianta organica di sette unità, che credo sarebbero in grado di rispondere al carico che si è venuto a determinare. Non c'è alcuna volontà di sopprimere nuove sedi di uffici di primo grado questo, tra l'altro, neanche è oggetto della riflessione della Commissione Vietti, la quale ha indicato alcuni criteri di carattere quantitativo (una corte d'appello per almeno un milione di abitanti). In verità, quello studio oggi è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura e non esprime ancora la volontà del Governo, che si formerà all'indomani dell'acquisizione del parere di tale organo. Per quanto riguarda Per quanto riguarda la questione della Corte di cassazione, non ho difficoltà a raccogliere l'invito che è stato rivolto. Il senatore Caliendo saprà che è stato costituito un gruppo un gruppo di studio tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della giustizia per affrontare la situazione della giustizia tributaria. Noi non escludiamo che l'esito di quel lavoro possa approdare alla proposta che lei ha avanzato e che potrebbe anche trovare un primo accoglimento in sede di approvazione del disegno di legge sulla giustizia civile, che dovrebbe essere sottoposto al più presto alla Commissione competente in questo ramo del Parlamento e che è già stato approvato Per quanto riguarda la questione della giustizia minorile, vorrei sottolineare come non ci si trovi di fronte a una volontà di sopprimere la giustizia giustizia minorile, ma di collocarla in un contesto più ampio, nel quale si affronti complessivamente il tema del funzionamento della famiglia e le eventuali patologie che possono avere riflessi sulla giurisdizione. Da questo punto di vista credo che questo intervento sia ancor più urgente all'indomani dell'intervento dell'intervento del legislatore che ha fortemente ridimensionato le competenze del tribunale dei minori e le ha frammentate tra una serie di soggetti diversi all'interno della giurisdizione. Il risultato è che ci sono alcuni uffici, senatrice Mussini, che davvero hanno pochissimo lavoro da fare (mi si consenta questa affermazione). Produrrò al più presto il carico di lavoro di alcuni tribunali dei minori. È un peccato, perché là si trovano, come lei ricordava, competenze di altissimo valore, che nel quadro della giurisdizione potrebbero dare una risposta davvero significativa. Il nostro intento è quello di costruire una struttura più ampia e robusta, che sia in grado di valorizzare il lavoro della cultura giuridica che ha sostenuto lo sviluppo dell'azione dei tribunali dei minori nel nostro Paese.

Signor Ministro, accolgo con favore le sue precisazioni e informazioni, soprattutto per quanto riguarda il tribunale e la procura di Vicenza. Naturalmente invito tutti noi a vigilare sulla corretta applicazione delle norme e, in particolare, sulla corretta applicazione delle norme concorsuali, perché effettivamente i posti vacanti che ci sono nel nostro sistema giustizia hanno bisogno di essere al più presto coperti.

dovrebbe essere fatto, possibilmente, prima che arrivi il personale delle Province, che avrà un altro tipo di qualificazione rispetto al personale la ringrazio per le delucidazioni che, però, non ci soddisfano. Il problema non è ampliare la pianta organica del tribunale di Reggio Calabria, che amplierà soltanto la percentuale dei posti scoperti, aumentando i posti che già sono scoperti. ci hanno riferito che c'è scopertura dei posti dell'ufficio del gip. Si richiedeva un intervento di carattere straordinario.

Proprio il tribunale di Reggio Calabria l'altro ieri è stato chiuso perché mancavano luce e acqua, a Catania manca l'aria condizionata e non si possono quasi tenere le udienze: se questa è la gestione passata dai Comuni al Ministero, siamo, purtroppo, in alto mare.

e la specializzazione, che non sono certamente garantibili se questi importanti servizi verranno assorbiti dai tribunali ordinari e se non sarà chiarita in modo estremamente trasparente e definitivo anche la funzione esclusiva

l'idea che si crea è che, in realtà, si voglia razionalizzare ed ottenere un risparmio su chi forse vale la pena tutelare per il futuro più di tanti altri. Ricordo che noi abbiamo il minor numero di detenuti nelle carceri minorili e il minor numero in Europa di recidive. Questo è un patrimonio da preservare.

per abolirlo, perché quando lei ha parlato degli accorpamenti dicendo che sarà il CSM a fare una proposta, è come se in una

abbiamo visto la sua straordinaria capacità anche nel riqualificare il personale e riteniamo che questo sia un punto cardine, perché pensiamo che

l'altro è estremamente delicato, anche in funzione della ripresa economica del nostro Paese. Tuttavia, come giustamente ha evidenziato in risposta alle nostre domande, sono i criteri che spesso dovrebbero essere

corte d'appello e il tribunale, a Potenza e a Matera. Credo che anche rispetto al criterio di favorire la giustizia nel miglior modo possibile,

GINETTI *(PD)*. Signor Ministro, in questi due anni di Governo e di attività parlamentare notevoli sono stati i risultati ottenuti sul fronte del sovraffollamento delle carceri,

che i provvedimenti citati abbiano terminato il loro effetto deflattivo e gli istituti sono tornati ad essere sovraffollati: contano oggi 54.000 detenuti e le Regioni più affollate sono Lombardia, Sicilia, Campania Pertanto, si chiede al Ministro cosa si intenda fare su questo fronte per alleggerire la situazione, anche perché essa coincide con un aumento degli eventi critici, legati anche a quella nuova modalità

l'attività di contrattazione con le organizzazioni sindacali per il riallineamento e il riordino del Corpo di polizia penitenziaria, che è chiamato ogni giorno, con spirito di servizio e sacrificio, a prestare la propria opera per garantire la sicurezza e l'ordine all'interno degli istituti. Infine, chiedo che cosa si intenda fare per dare, dopo quarant'anni, concreta attuazione ad un ordinamento specifico per i minori, visto che in questi quarant'anni con interventi sporadici e non organici. In ultimo, chiedo che cosa si intenda fare per la qualità edilizia degli istituti carcerari (in particolare sto pensando all'istituto di Sollicciano, segnalato anche con un ordine del giorno specifico dal Consiglio comunale da Firenze).

Lei sa meglio di me che nella passata legislatura finalmente è stato avviato un processo di realizzazione di 4.250 posti detenuti, che sono stati in parte ultimati in questa legislatura, mentre altri interventi sono stati operati dal suo Governo, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero dei detenuti. Probabilmente dobbiamo proseguire anche nella costruzione di ulteriori posti detenuti. Il secondo aspetto

Smuraglia; però è ridotto quasi a 4 milioni quanto è destinato al lavoro all'interno delle carceri. Credo sia necessario un ulteriore accorgimento: utilizzare i detenuti anche per lavori diversi all'interno delle carceri, fossero anche di piccola manutenzione della struttura carceraria, per la finalità che dobbiamo dare alla pena e nella consapevolezza che il lavoro può dare al detenuto una speranza e la certezza di non recidiva. Per questa ragione credo che dovremmo tentare

Signor Ministro, la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno definito il lavoro dei detenuti un diritto fondamentale. Eppure nel nostro Paese sono solo un esiguo numero i detenuti che godono di tale diritto, diversamente da quanto accade in moltissimi altri Stati europei e naturalmente negli Stati Uniti. I vantaggi del lavoro in carcere sono molteplici. Si offre ai detenuti la possibilità di acquisire delle competenze spendibili nel mercato del lavoro, a conclusione dell'espiazione della pena. Si agevola inoltre il reinserimento dei detenuti nella società, con evidente diminuzione della possibilità di tornare a delinquere successivamente, come dimostrano peraltro numerose statistiche, che vedono un'apprezzabile riduzione del tasso di recidiva tra i detenuti lavoratori. Non ultimo, il lavoro avrebbe indubbiamente effetti positivi anche sullo stato psicologico delle persone che sono costrette nelle carceri. Attualmente non solo lavorano pochissimi detenuti, peraltro a rotazione e in modo discontinuo, ma appena l'1 per cento di loro si occupa di manutenzione ordinaria dei fabbricati, fronte sul quale l'amministrazione è costretta a spendere ingenti risorse pubbliche in appalti esterni o, più frequentemente, a rinunciare all'attività manutentiva per mancanza di risorse. Alla luce di quanto esposto si chiede, signor Ministro, quali siano le motivazioni per cui nel nostro Paese il numero di lavoratori detenuti continua ad essere ridottissimo, nonostante tutti i vantaggi che abbiamo esposto, e se e con quali modalità intenda procedere, limitatamente alle sue competenze, nel dare piena applicazione al lavoro in carcere in quanto componente essenziale del processo di rieducazione garantito dalla Costituzione. *(Misto)*. Signor Ministro, farò questo passaggio logico. Il sovraffollamento carcerario sicuramente è uno dei nodi critici del sistema giudiziario del nostro Paese. Abbiamo assistito ad una flessione al ribasso, che è stata legata anche a delle modifiche del sistema di repressione dei reati. I più recenti provvedimenti posti in essere per rimediare a questa situazione hanno contribuito ad un incremento notevole del numero di condannati, cui l'ordinamento, in presenza di determinati presupposti, riconosce la possibilità di espiare la pena irrogata con modalità diverse rispetto al regime detentivo, il che ha permesso sicuramente di ridurre la pressione e il sovraffollamento carcerario.

introdotti dal legislatore per attenuare il sovraffollamento carcerario. Ora, su tutto il territorio nazionale si lamenta una situazione di gravissimo disagio,

quanto riguarda le città di Bologna e di Modena. Voglio ricordare però che la specifica realtà territoriale del distretto di Bologna è particolarmente in crisi. Le ho inviato un'interrogazione che entra più nel dettaglio di questa realtà e alla quale spero che lei voglia dare prontamente risposta.

Signor Presidente, mi rifaccio a quanto la collega Ginetti in via generale ha affermato parlando del sovraffollamento. Io scendo nel particolare, perché condivido e sottoscrivo il suo intervento, per sapere perché non si costruiscono le carceri. Nel 2010 è stato fatto un piano carcerario dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi in cui si prevedeva la realizzazione di diverse

Eppure si sono già spesi oltre 2 milioni di euro che il Ministero dovrà pagare. Si chiede pertanto di sapere se vi sia intenzione di procedere a tale ampliamento e di sollecitare la firma del contratto, visto che i documenti sono già stati tutti richiesti, e se, trattandosi di un appalto pubblico

I detenuti denunciano da tempo il grave stato di decadimento e di pressoché assente manutenzione di diverse sezioni; i locali cucina e il locale docce del vecchio padiglione versano in condizioni igienico-sanitarie particolarmente critiche, con la presenza di muffe,

da un compagno di cella (si tratta nello specifico di uno straniero). Il signor Andrea Gambis, sezione 1, non può lavarsi autonomamente perché il locale docce è sprovvisto dei corrimano e degli ausili necessari ai portatori di disabilità. Altrettanto gravi sono le condizioni di vita della polizia penitenziaria, per via dell'organico insufficiente e di turni di lavoro straordinario sistematici, che costringono il personale a fronteggiare da soli situazioni potenzialmente potenzialmente pericolose, quali aggressioni, tentativi di suicidio o atti di autolesionismo. Inoltre, l'amministrazione dovrà gestire l'imminente apertura di un polo psichiatrico, richiedente personale medico-sanitario ad oggi non individuato. Ricordo, infine, che gli alloggi dove il personale di polizia è costretto a risiedere, in quanto la maggior parte è fuori sede, dietro pagamento di un contributo mensile, sono estremamente angusti, insalubri a causa delle infiltrazioni, poco funzionali e con bagni inadeguati. Mi permetto, quindi, di chiederle se non sia possibile provvedere a un rimodernamento delle carceri esistenti a livello nazionale e a una contestuale implementazione dei programmi di formazione dei detenuti, per migliorare le loro condizioni in carcere,

stranieri, inneggiando ad Allah e all'ISIS, hanno interamente sfasciato una sezione del carcere, costringendo all'intervento della polizia penitenziaria in tenuta antisommossa.

(tra l'altro, questi detenuti beneficiano del regime aperto, come coloro che hanno una buona condotta). Per questa ragione, anche i vari agenti del Sappe hanno denunciato i fatti, lamentando in particolare la situazione riguardante la dirigenza.

in ossequio al dettato normativo, il regime speciale prevede la custodia dei detenuti all'interno di sezioni speciali sorvegliate da personale di polizia penitenziaria specializzato che dovrebbe essere, oltre che adeguatamente formato, proporzionato nei numeri alla popolazione detenuta destinataria di tale regime. In realtà, non so se a lei è noto, ma l'unica struttura che allo stato risulta idonea al perseguimento dei fini previsti dall'articolo 41-*bis* della legge penitenziaria risulta essere la casa circondariale di Sassari.

allora di sapere se costoro possono dedicarsi all'attività per la quale vengono addestrati? Esiste una predefinita pianta organica dei reparti in argomento e, in caso positivo, è rispettata? Esistono dei corsi di formazione/aggiornamento specificamente dedicati ai reparti specializzati e, in caso positivo, con quale frequenza sono svolti? In altri termini, vi è un coerente programma di selezione, formazione e integrazione del personale specializzato che sia confacente alle esigenze sottese allo speciale Inoltre, in tema di prevenzione, sarebbe interessante sapere se l'assegnazione dei compiti precipuamente previsti dalla norma di riferimento (controllo della corrispondenza, controllo dei colloqui, ascolto delle telefonate) sia lasciata al caso ovvero all'iniziativa e volontà dei singoli direttori di istituto, piuttosto che frutto di criteri prestabiliti e omogenei per tutti gli istituti. Presidente, una considerazione di carattere generale dalla quale vorrei partire è questa. Quando si è insediato questo Governo il tasso di sovraffollamento

sovraffollamento, perché dà conto di un lavoro che è stato compiuto. I detenuti erano 60.971, a fronte di circa 44.000 posti disponibili. Attualmente i detenuti sono circa 54.070, a fronte di 49.701 posti disponibili. Ma non è tanto questo il dato sufficiente a dare una risposta. Piuttosto, io vorrei partire da una considerazione rispetto ad una affermazione che ho sentito fare fare anche in quest'Aula in altre occasioni, cioè che la diminuzione del sovraffollamento avrebbe comportato una ripercussione sulla dimensione della sicurezza. Vorrei ricordare come, a fronte dei 21.000 soggetti ammessi a misure alternative al carcere del dicembre del 2010 (che prendo sempre come anno di riferimento e punta massima della crisi),

deve essere mirato a un utilizzo ulteriore delle pene alternative. In questo senso abbiamo potenziato - e stiamo ulteriormente lavorando in questa direzione - gli uffici di esecuzione penale esterna, istituendo anche un Dipartimento all'interno del Ministero che si occupa congiuntamente di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, perché la messa alla prova non casualmente è stata elaborata e sperimentata prima nell'ambito del minorile e poi è stata trasposta dal legislatore anche nell'ambito degli adulti. quindi una realtà nella quale si può sviluppare pienamente il concetto di esercizio delle pene alternative e delle cosiddette sanzioni di comunità. L'altra linea sulla quale ci vogliamo muovere e ci stiamo muovendo è quella del rimpatrio dei detenuti stranieri. di questo tema si parla da tantissimo tempo, ma con mia somma sorpresa quando mi sono insediato al Ministero ho scoperto, per esempio, che non esisteva un trattato di estradizione con una Nazione che contribuisce a determinare una quota significativa di detenuti, cioè il Marocco. Il mese successivo al mio insediamento mi sono recato a Rabat per sottoscrivere questo accordo, che ancora naturalmente attende un'esecuzione ma che è il presupposto per questo tipo di attività. Contemporaneamente abbiamo lavorato sul fronte dei Paesi con i quali erano consolidati dei rapporti per aumentare il flusso del rientro dei detenuti stranieri, in particolar modo con l'Albania e con la Romania. Credo che alcuni segnali siano arrivati e alcuni numeri ci confortano in questo senso, ma non siamo ancora davvero all'altezza delle aspettative che abbiamo. In terzo luogo c'è un altro lavoro che abbiamo predisposto: ho firmato con quasi tutte le Regioni italiane dei protocolli per l'esecuzione penale per i tossicodipendenti, affinché sia pienamente rispettata l'indicazione, contenuta tra l'altro nella legge Fini-Giovanardi, che consente l'esecuzione di pene alternative in comunità quando appunto ci siano determinati requisiti, esecuzione che oggi non è compiutamente realizzata perché molte Regioni non mettono a disposizione i posti necessari e quindi il magistrato di sorveglianza si trova nella condizione di non poter assegnare la pena alternativa. Detto questo abbiamo anche lavorato sul fronte dell'aumento della disponibilità di posti e lo dicono i numeri. Lo abbiamo fatto portando a compimento alcune opere che erano già *in itinere*. Ho inaugurato il carcere di Rovigo ed entro la fine di luglio sarà inaugurato il carcere di Vicenza. Abbiamo utilizzato, via via che venivano chiusi, gli ospedali psichiatrici giudiziari - che sono a tutti gli effetti strutture funzionali alla detenzione - e abbiamo ipotizzato ulteriori interventi, meno di quelli che erano previsti nel cosiddetto piano carceri varato dal governo Berlusconi. Riteniamo, infatti, che un adeguato sviluppo delle pene alternative possa consentire anche di avere obiettivi meno alti rispetto all'insieme dei posti disponibili; il sistema si dovrebbe assestare intorno ai 53.000-54.000 detenuti, numero che attualmente risulta. Naturalmente in questo dato c'era inevitabilmente un elemento di alea, perché non sapevamo se i conti potevano tornare, anche perché le variabili sono moltissime. Non si tratta soltanto di capire quali sono in media i reati perseguiti in una fase piuttosto che in un'altra; abbiamo visto in alcune occasioni picchi e crescite non facilmente prevedibili perché in mezzo c'è poi l'attività di carattere processuale, con tutte le sue velocità e le sue lentezze, a seconda del tipo di reato contestato. Tuttavia, iniziamo a ritenere che l'assestamento ci sia, perché dopo un aumento che negli ultimi sei mesi era tornato a caratterizzare il numero dei detenuti - che erano passati da sotto i 53.000 ai 54.000 di questo mese - questo è il primo mese, se nel quale i detenuti sono tornati a scendere, seppur di poco. Ad ogni modo, questo mese c'è stata una diminuzione, che riteniamo possa voler dire che ci siamo avvicinati al punto di equilibrio. Ciò significa che non dobbiamo più fare carceri? No, in alcune realtà avevamo pensato si potesse evitare la realizzazione di alcune carceri, ma bisogna considerare il tasso di sovraffollamento Regione per Regione perché il punto fondamentale è che molti detenuti hanno diritto ad una garanzia del legame territoriale con alcune realtà. Ebbene, questo

su quell'episodio sta indagando ancora oggi la procura distrettuale di Bologna. Esso Esso è stato contenuto rapidamente dalla direzione della casa circondariale; infatti, non sono rimasti feriti né agenti né detenuti e non è stato nemmeno necessario chiudere la sezione detentiva. Quanto al rilievo mosso all'applicazione del regime aperto ai detenuti stranieri di religione islamica protagonisti dell'episodio, si evidenzia che la direzione ha immediatamente assunto tutte le misure e che il regime di sorveglianza particolare non è stato applicato perché per uno dei detenuti stranieri era in corso la procedura di espulsione dal territorio dello Stato, che è stata immediatamente attuata, e per un altro a causa delle sue gravi condizioni psichiatriche che lo sconsigliavano. Per quanto riguarda il tema del lavoro, vorrei riferire come abbiamo svolto una significativa azione che ha visto, nelle relazioni che in questi anni abbiamo consegnato al Parlamento, in questi anni abbiamo consegnato al Parlamento, crescere costantemente il lavoro all'interno delle carceri, seppure di poco. Nel corso del 2015 sono stati finanziati dalla Cassa delle ammende 267 progetti, mentre dall'inizio del 2016 sono stati già presentati 148 progetti dello dello stesso genere. Cosa credo si debba e si possa ancora fare? Noi abbiamo fatto un lavoro per realizzare uno sgravio anche in esecuzione della legge Smuraglia. Devo dire che le risposte imprenditoriali sono state contenute, tanto che noi stiamo pensando di istituire un soggetto che in modo permanente svolga un'attività di promozione dell'utilizzo del lavoro all'interno del carcere, che, come tutti gli altri tipi di lavoro, funziona se si

Io non ho tenuto conto di quell'indicazione, ma devo dire che a contrastare quella polemica mi sarebbe piaciuto ci fossero più forze politiche, perché credo che credo che vadano fatte delle battaglie anche quando, come in questo caso, non danno grande popolarità. Ritengo che questo sia un dato che ci dovremo ricordare, perché per proseguire questo lavoro noi incontreremo molti altri ostacoli di questa natura, cioè di carattere culturale e di argomentazione populista, che però credo debbano essere battuti con le argomentazioni che lei ha sottoposto a questa discussione e che io condivido pienamente. Vorrei poi sottolineare - lo dico anche sottolineare - lo dico anche perché in quest'Aula sono presenti tutte le forze politiche e in questo possono farsi parte attiva - come ci sia da incoraggiare ancora di più l'utilizzo del lavoro dei detenuti nell'ambito della convenzione firmata con l'Associazione nazionale Comuni italiani,

Per quanto riguarda il tema dal carcere di Sollicciano, posto dalla senatrice Ginetti, vorrei riferire che la situazione è nettamente migliorata sul versante della struttura, delle condizioni di vita dei detenuti e con specifico riferimento al potenziamento delle attività trattamentali, grazie alle azioni che abbiamo intrapreso nel corso degli ultimi mesi, come ha riconosciuto anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. Questi primi risultati ci incoraggiano a proseguire un'opera che naturalmente deve essere portata a compimento. Vorrei poi riprendere un'altra questione sollevata, cioè come riteniamo di poter dare una risposta al al ruolo fondamentale svolto dalla polizia penitenziaria. Io mi onoro di essere il primo Ministro ad aver agito nella direzione dell'allineamento delle carriere del Corpo della polizia penitenziaria penitenziaria con gli altri Corpi. Come lei sa, però, senatrice Ginetti, il passaggio necessario è quello del raccordo con le altre forze di polizia, secondo quanto contenuto all'interno

Ci sono - è vero - attività di formazione per chi svolge funzioni di carattere speciale, che hanno una cadenza periodica, della quale onestamente non le saprei riferire

così come credo risponderebbero quasi tutti i miei colleghi che hanno un portafoglio e che oggettivamente scontano il fatto che in tutta la pubblica amministrazione c'è stato un blocco pluriennale Nell'ambito del decreto sicurezza c'è stata una previsione per l'assunzione di un numero aggiuntivo di agenti di polizia penitenziaria. Noi auspichiamo che queste Noi auspichiamo che queste assunzioni possano essere realizzate al più presto e in questo senso mi sto già facendo parte attiva.

fino a 49.701 per i detenuti, sia per questa linea di indirizzo nel rafforzamento dell'esecuzione penale esterna, cui naturalmente auspichiamo possa conseguire anche il rafforzamento degli uffici per l'esecuzione esterna, nelle diverse figure professionali comunque mancanti. La ringrazio per l'attenzione che continua a riservare anche ai fini di un'accelerazione per quanto riguarda la valorizzazione del Corpo di polizia penitenziaria e il riallineamento.

L'unica cosa su cui non siamo d'accordo è che io ritengo necessaria almeno la realizzazione di altri 3.000 posti detenuti, per rendere ormai stabile la compatibilità tra posti disponibili e numero dei detenuti.

per legge ma immediatamente reso nullo da un successivo concorso a distanza di pochi mesi dall'approvazione della legge. Signor Presidente, signor Ministro, noi non saremo soddisfatti fino a quando non riusciremo a ribaltare la percentuale di detenuti che lavorano e di detenuti che rimangono tutto il giorno nell'ozio delle loro celle. Partiamo almeno dalla manutenzione ordinaria degli istituti penitenziari e dei fabbricati: sarebbe già una buona partenza e costituirebbe un passo di civiltà (uso questo termine).

Signor Ministro, lei non mi ha risposto, ma la ringrazio lo stesso perché è venuto e ha risposto ad altre domande, anche se non a questa, e ha sicuramente fatto molto di più

sarà contemporaneamente affrontato anche tutto quel mondo variegato, fatto di responsabilità condivise e di competenze varie ed estese, contenuto nelle misure - che io condivido - che puntano di più sulla riabilitazione e sull'integrazione.

Signor Ministro, mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Sono soddisfatto per i temi generali, che ha affrontato molto bene e che effettivamente danno un quadro in miglioramento della situazione: innegabili i dati numerici che lei ha fornito e i tre punti che lei ha ben sviluppato sulle pene alternative, sul rimpatrio dei detenuti stranieri (obiettivi assolutamente da perseguire) e sull'attenzione alla tossicodipendenza.

Lei certamente saprà che non sono uno che ha condiviso molto delle riforme che il suo Governo ha fatto; anzi, per la stragrande maggioranza non le condivido, però le darei il suggerimento di provare a fare un'ulteriore riforma nel sistema penitenziario guardando soprattutto a chi deve amministrare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria evitando per il prossimo futuro